Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri sera, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 28 maggio. Nel comune intento di concludere l'esame del disegno di legge collegato su internazionalizzazione imprese ed energia entro la giornata di domani, si è proceduto ad un'integrazione dei tempi a disposizione dei Gruppi che li hanno esauriti, attribuendo al Partito Democratico e al Popolo della Libertà 40 minuti ciascuno. Nella rimanente parte di questa settimana, che prevede votazioni anche nel pomeriggio di domani, saranno inoltre discusse - se possibile - le mozioni Sbarbati e Possa, sulla promozione della cultura, e Bianchi, sulla Carta europea dei diritti del malato, nonché le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione. Diversamente, tali argomenti saranno trattati la prossima settimana. La discussione del disegno di legge di conversione del decreto‑legge sul terremoto in Abruzzo, già prevista per la giornata di domani, avrà invece inizio a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 19 maggio, al fine di assicurare un ampio lavoro istruttorio alla Commissione competente. Nella seduta pomeridiana di giovedì 21 maggio si svolgeranno interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151*‑bis* del Regolamento. Nel corso di tale giornata sarà inoltre ricordata la figura di Massimo D'Antona nel decimo anniversario della sua morte. in vista della sospensione dei lavori prima della tornata elettorale del 6-7 giugno, l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di lunedì 25 maggio, per l'esame - fino alla seduta pomeridiana di mercoledì 27 degli argomenti non conclusi in precedenza e del disegno di legge collegato su sviluppo economico, semplificazione e processo civile. La seduta antimeridiana di giovedì 28 maggio riguarderà il sindacato ispettivo. Nella riunione della Conferenza dei Capigruppo da convocarsi la prossima settimana saranno poi presi in considerazioni gli ulteriori argomenti sollecitati dai Gruppi. È stato infine stabilito che l'Assemblea non terrà seduta nella settimana antecedente le elezioni europee e amministrative del 6-7 giugno. L'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 9 giugno secondo il calendario che sarà successivamente definito. Le Commissioni potranno convocarsi in relazione ad esigenze dei rispettivi programmi dei lavori.

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 2.250, 1.300 (testo 3), 16.500, 18.750, 18.0.300/1 (testo 2)

33-*quinquies*.304. Esprime poi parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 6.301 (testo 2), 32-*bis*.0.301, 32-bis.0.302,

quanto meno distratta, in una seduta molto particolare, caratterizzata da ripetuta mancanza del numero legale e

che le Regioni dovrebbero continuare ad essere protagoniste di un fenomeno che riguarda in modo diretto le loro coste.

pericoloso, molto rischioso per la città di Venezia. Ed è per questo motivo che oggi lo Stato italiano sta già spendendo 5 miliardi di euro per difendere la città di Venezia. Il fenomeno della subsidenza è poco prevedibile,

seguito all'estrazione di un quantitativo così consistente di gas. La prova dell'esistenza di questo rischio è data dal fatto che è stata proibita, dopo essere stata avviata, l'estrazione del gas nell'area

Debbo dire, vice ministro Urso, che non avrei difficoltà, ancora una volta, anche contro le mie personali opinioni, a dare l'assenso ad una norma che è visibilmente nell'interesse dell'ENI, se se il Governo accettasse di modificare questa particolare previsione, introducendo la garanzia di una valutazione tecnica indipendente internazionale.

abbiamo trattato un argomento di grande interesse, quello della subsidenza, che ha provocato in passato e sta provocando confronti e scontri a livello regionale e anche interregionale; basta immaginare quello che sta facendo la Croazia nella stessa area.

la mancanza di paletti necessari a garantire che il tutto sia effettuato secondo il rispetto di certe procedure. Basterebbe verificare giustamente, la valutazione di impatto ambientale e la condivisione con le autorità locali; c'è comunque l'assoggettabilità, nel caso del comma

che delega il Governo a predisporre la normativa per il riassetto del settore e per l'individuazione della localizzazione dei siti nucleari. Oggi, uno dei più importanti e diffusi quotidiani nazionali presenta una possibile mappa di localizzazione di questi siti nucleari:

anni '70. Si può immaginare come questa possibile - o improbabile: dipende dai punti di vista - localizzazione crei già in queste ore allarme e preoccupazione, a conferma - mi rivolgo al viceministro Urso che so essere sensibile a questi temi - della validità di una delle questioni che abbiamo posto ieri: la necessità cioè che questo intervento del Governo prevedesse un'intesa con gli enti locali e le Regioni. Ma i nostri emendamenti in questo senso, purtroppo, non sono stati accolti

perché si ragioni in maniera seria e approfondita, non inseguendo improbabili previsioni giornalistiche o studi di molti anni addietro, che il Governo smentisca, magari già in quest'Aula oggi stesso, che questi siti siano attuali

Mi auguro che nella realizzazione e nell'attuazione dello stesso si possa porre rimedio e coinvolgere pienamente le istituzioni e le Regioni.

Ovviamente, a questo si arriverà secondo quanto previsto dalla legge che stiamo per approvare in questa sede, che è molto rispettosa delle decisioni degli enti locali e che terrà conto appieno di tutte le normative sulla sicurezza che sono previste dall'Unione europea. Si tratta dunque di un articolo privo di fondamento. Credo sia stato fatto esclusivamente al fine di creare un clima negativo nei confronti di una legge che invece il Paese aspetta da tempo. Non a caso cita città e luoghi in cui si voterà tra pochi giorni. Quindi, ripeto, è di natura meramente elettorale e assolutamente infondato.

**Il Senato non approva.**

copertura, assumendo che non si dovessero determinare incrementi di costi per mettere in campo iniziative tese a meglio definire le modalità di tutela della salute dei cittadini e di salvaguardia dell'ambiente in relazione alla reintroduzione del nucleare nel nostro Paese. l'emendamento in esame si mettono a disposizione 3 milioni di euro per un'attività di analisi e valutazione statistica nel settore energetico per acquisire dati già oggi disponibili per tutti quindi, a maggior ragione, per gli uffici del Governo che contribuiscono a raccoglierli, classificarli e valutarli.

La motivazione alla base dell'emendamento, che è comprensibile e condivisa, può essere sintetizzata nel principio della diminuzione della sanzione (allora prevista in un importo

stabilendo che nei piccoli bacini, dove sopravvivono vecchi consorzi e vecchie aziende municipalizzate, le sanzioni fossero paragonate anche al volume

sanzionatori leggeri mentre ai grandi distributori di energia si possono irrogare anche sanzioni più pesanti.

significative di questo articolo che riguarda il funzionamento dell'Agenzia sulla sicurezza nucleare, che dovrebbe vigilare appunto sulla sicurezza degli impianti vecchi, nuovi, sulla sicurezza delle attività anche di *decommissioning* delle centrali e di smaltimento delle scorie.

una modifica linguistica, ma in realtà sfugge francamente come si possa chiedere ad un organismo, qualunque esso sia, di garantire la sicurezza nucleare; ad un organismo pubblico o privato di garantire la sicurezza antisismica. Si tratta di un'espressione che tradisce la visione un po' fideistica e ideologica che il Governo e la maggioranza hanno di questo ritorno all'energia nucleare. Chiediamo pertanto che si utilizzi un'espressione un po' più appropriata e razionale come quella per cui l'Agenzia deve vigilare sulla sicurezza nucleare, che è il massimo che realisticamente può fare. L'emendamento 17.23, che riguarda sempre il comma 4, chiede che l'Agenzia sia tenuta a presentare annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare e che tale relazione debba essere discussa e approvata dal Parlamento stesso. In questo caso crediamo, caso crediamo, attraverso questa proposta di modifica, di rendere più trasparenti i meccanismi di informazione e di accesso all'informazione per quanto riguarda il nucleare e soprattutto l'eventuale ritorno alla realizzazione centrali nucleari. Riteniamo che in questo scenario si debba fare tutto lo sforzo possibile perché il Parlamento sia coinvolto a pieno titolo e nella pienezza delle delle sue funzioni nel controllo di queste informazioni. L'emendamento 17.37 è un'altra proposta importante la quale si chiede di inserire dopo il comma 5 il comma 5*-bis*, nel quale si specifichi che l'Agenzia sulla sicurezza nucleare debba avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle Agenzie regionali per l'ambiente. Queste ultime sono un sistema, come si sa, esistente da tempo, in alcuni casi anche molto ben funzionante; un sistema che già oggi ha in sé competenze, risorse umane, che riguardano in particolare il controllo della radioattività. Noi crediamo che in una materia concorrente, come quella della produzione e distribuzione di energia, sia necessario e decisivo che l'Agenzia nasca e funzioni in uno stretto rapporto con le Regioni, da una parte, e con il sistema delle Agenzie regionali per l'ambiente, dall'altra.

di nomina e la composizione degli organismi dell'Agenzia. Attraverso questa proposta di riscrittura del comma 6 vogliamo fissare due princìpi che riteniamo irrinunciabili: il primo è quello per cui tra i quattro membri dell'organo collegiale che guida l'Agenzia, uno debba essere indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano proprio perché stiamo parlando di una materia costituzionalmente concorrente tra Stato e Regioni. Quindi l'organismo che presiede alla vigilanza sulla produzione di energia nucleare non può non prevedere la presenza al suo interno del sistema dei governi regionali. L'altro principio che vogliamo affermare riguarda l'esigenza vogliamo affermare riguarda l'esigenza che l'Agenzia sulla sicurezza nucleare non diventi, come purtroppo sembra essere l'intenzione del Governo e della maggioranza, un organismo che risponde a criteri di parte, di schieramento. Chiediamo che la nomina dei membri dell'organismo collegiale che guida l'Agenzia debba sottostare ad un parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, proprio per garantire a tutti cittadini che l'Agenzia sulla sicurezza nucleare agisca secondo criteri di rappresentanza dell'interesse generale e non secondo criteri di rappresentanza dell'interesse politico della maggioranza che di volta in volta governa il Paese. Oggi è il centrodestra, ma - a prescindere da questa circostanza - la essere il *dominus* della competizione e quindi anche degli orientamenti di lavoro e di attività dell'Agenzia sulla sicurezza nucleare. L'ultimo emendamento che vorrei brevemente illustrare è il 17.58. caso ricorre con grande evidenza la tentazione da parte del Governo e della maggioranza di

debba garantire e assicurare, nei limiti del possibile, lo svolgimento dei propri compiti in modo davvero autenticamente indipendente e davvero autenticamente terzo.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta Esprime poi parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alle seguenti condizioni: - che all'emendamento 6.301 (testo 2) il secondo periodo sia cosi sostituito: "Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2009 quanto a euro 500.000 l'accantonamento dei Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento del Ministero dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze."; che all'emendamento 1.300 (testo 3) venga soppressa la lettera *c)*. Esprime poi parere di semplice contrarietà sulla lettera *d)* dell'emendamento 1.300 (testo 3). Esprime infine parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti

parere conforme al relatore su tutti gli emendamenti,

La posizione del Governo sembra essere contraria all'emendamento 17.25, che dispone che l'Agenzia per la sicurezza nucleare operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Sarebbe veramente strano che questo emendamento venisse bocciato; sarebbe veramente grave che si lasciasse soltanto lontanamente ipotizzare che l'Agenzia per la sicurezza nucleare possa agire in condizioni di non indipendenza e di non piena autonomia di giudizio e di valutazione.

ci siamo permessi di proporre una modalità di nomina dei membri che costituiscono quell'organo attraverso le procedure più garantiste, solo comportano una evidenza pubblica per l'acquisizione dell'interesse degli esperti a parteciparvi una validazione e una valutazione delle competenze scientifiche, tecniche e professionali dei candidati,

e che può essere risolto in coerenza con la civiltà giuridica che nel nostro Paese è già operativa, con risultati più che soddisfacenti.

importante che questa Agenzia possa relazionare ogni anno sui propri lavori: quindi il Gruppo dell'Italia dei Valori darà un voto favorevole a questo emendamento.

indicato in questo disegno di legge di un ritorno dell'Italia all'energia nucleare, è assolutamente condivisibile, talmente condivisibile che l'Agenzia è frutto di proposte che alla Camera sono state avanzate dal Partito Democratico. Nella iniziale formulazione del disegno di legge in discussione non era infatti

di riempire di contenuti appropriati le funzioni, i criteri di costituzione e la composizione degli organismi collegiali di direzione dell'Agenzia, testimonino l'approccio

delle garanzie indispensabili per una istituzione i cui compiti sono così delicati

delle maggioranze che di volta in volta governano il nostro Paese. Poche settimane fa, nel suo discorso di commiato dall'Italia, l'ex ambasciatore degli Stati Uniti, Spogli,

fare di tutto perché non sia una scelta di maggioranza. Ai criteri di indipendenza dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (altrettanto importanti rispetto

l'Agenzia sia tenuta a presentare una relazione annuale al Parlamento sulla sua attività e sul suo funzionamento. Evidentemente, si è preoccupati persino di questo piccolo margine di accessibilità alle informazioni da parte del massimo organo rappresentativo della sovranità dei cittadini del nostro Paese. Nei suoi criteri di funzionamento e composizione, l'Agenzia non risponde nemmeno - io credo - al contenuto dell'articolo 117 della Costituzione, che colloca la produzione e la distribuzione di energia tra le materie di tra Stato e Regioni. Noi abbiamo chiesto, ad esempio, che uno dei membri dell'organismo collegiale che dirigerà l'Agenzia per la sicurezza nucleare sia espresso dalla Conferenza unificata Stato-Regioni: questa proposta è stata respinta, così come sono state rigettate altre proposte analoghe. Credo che anche in questo risieda uno dei limiti, non solo dell'articolo 17, ma di gran parte del disegno di legge

una sorta di imballaggio abbastanza innocuo dal punto di vista della libertà di scelta senza controlli che il Governo vuole prendersi in relazione alla nuova stagione del nucleare che ha intenzione di aprire in Italia. Verrebbero così sostanzialmente contraddette le ragioni stesse per cui sarebbe necessario, utile e decisivo che in Italia, da oggi in avanti, operasse un'Agenzia per la sicurezza nucleare davvero forte nelle sue competenze e nella sua disponibilità di risorse umane ed economiche, indipendente e terza. Per queste ragioni, il Gruppo del Partito Democratico voterà contro l'articolo 17.

Con il primo chiediamo di introdurre una gradualità di attuazione della norma di cui all'articolo 18 per condizionarla al raggiungimento di un sufficiente grado di concorrenza nel mercato del gas. Proponiamo, quindi, di affidare al Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la determinazione di tempi e gradi successivi di apertura. Questo perché ancora il mercato del gas non è effettivamente liberalizzato; l'operatore dominante controlla la gran parte dell'offerta e delle infrastrutture di accesso. Sarebbe inutile applicare il modello di mercato elettrico, come auspicato dall'articolo 18, a quello del gas con gestione affidata alla borsa del gas e quindi fornitura dei clienti domestici da parte dell'acquirente unico perché, in questo caso, l'acquirente unico non sarebbe in grado di contrattare veramente con l'operatore dominante - quindi principalmente con l'ENI - ma si limiterebbe ad acquistare il gas a prezzi non reali, forse anche superiori a quelli in questo momento fissati dall'Autorità.

non sono stati in grado di innescare un effettivo processo concorrenziale che effettivamente favorisse il consumatore finale. A questo punto, vorremmo che fosse previsto, ove si volesse effettivamente raggiungere una concorrenza nei settori della vendita dell'energia, la netta separazione tra le diverse attività che rientrano nel processo di distribuzione e fornitura di energia e non solo l'introduzione di limiti alla possibilità di integrazione verticale tra le aziende del settore.

Si corre il rischio che il prezzo venga fissato sempre dall'ENI e che anche questo acquirente unico, sulla falsariga di quanto avviene per la borsa elettrica, si limiti, di fatto, a rifornirsi dall'ENI con nessuna possibilità negoziale. Il risultato sarebbe che l'acquirente unico acquisterebbe il gas non a prezzi di mercato, quindi superiori a quelli oggi determinati dall'Autorità per il gas e per l'energia. Per scongiurare questo scenario per le famiglie, occorre attribuire un chiaro potere al Ministro competente di assumere misure idonee a rendere il mercato più competitivo e di dettare conseguentemente i tempi della riforma.

l'incentivo, è necessario in particolare: prevedere l'incentivo soltanto per gli impianti destinati a coprire l'autoconsumo delle piccole imprese e dei clienti domestici, con impianti integrati negli edifici ed escludendo comunque l'installazione a terra;

L'emendamento 18.57 è volto all'estensione degli incentivi CIP6 anche ai teromovalorizzatori, laddove siano limitati alla frazione biodegradabile dei rifiuti inceneriti, che sarebbero altrimenti destinati a finire in discarica. Si deve esprimere invece assoluta contrarietà all'estensione degli incentivi anche alla quota non biodegradabile - o potenzialmente riciclabile - del rifiuto, in quanto si produrrebbe l'effetto di rendere più conveniente bruciare i rifiuti piuttosto che provvedere alla raccolta differenziata.

sono stati abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 ed i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, che prevedevano l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica ai contratti di compravendita e di locazione, insieme alla sanzione di "nullità relativa" di detti contratti, in caso di mancata allegazione di detta certificazione. Con l'emendamento 18.54 intendiamo invece ripristinare tale previsione, in mancanza della quale non vi sarebbe trasparenza nel mercato immobiliare perché non si consentirebbe ai cittadini che si apprestano ad acquistare o affittare un'abitazione, di essere al corrente dei costi energetici di gestione della casa e, soprattutto, di conoscere quali interventi effettuare per migliorare l'efficienza energetica delle unità immobiliari.

si gioca la presenza in Italia dei settori produttivi dell'alluminio, dello zinco e del piombo primari, i cosiddetti metalli non ferrosi.

elettrico competitivo con la fine delle tariffe elettriche agevolate, perché, così com'è scritta, la norma durerebbe solo pochi mesi, quindi per un periodo totalmente ininfluente e impeditivo dello sviluppo di qualsiasi piano industriale di mantenimento.

che costituisce un sistema di distretto di produzione energetica ed industriale insieme, si applicano le norme sulle reti interne di utenza come previste, su proposta del Governo, nella presente legge.

invece il Parlamento a produrre dei testi che sono stati letteralmente smontati e bloccati dall'Unione europea. Voglio dirle che se ciò accadesse un'altra volta il Governo non potrebbe essere assolto con la motivazione di non avere compreso il fatto, visto che noi abbiamo contribuito a spiegare.

che preveda un contemperamento tra l'effettivo costo evitato di combustibile, relativo alla nuova capacità produttiva realizzabile al momento dell'avvio della singola iniziativa avente diritto alla numerazione di cui al CIP n. 6/92, ed il rendimento di conversione

Presidente, l'emendamento 18.0.11 tende ad agevolare

propongo di sostituire le parole da "agli impianti" fino a "potenziamento" con le seguenti: «alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,

In occasione della Conferenza dei Capigruppo di ieri, tenuto conto del fatto che alcuni Gruppi avevano già esaurito i tempi loro assegnati, la Presidenza ha proceduto

ai Gruppi dei tempi residui, che tengono conto già della nuova attribuzione degli ulteriori spazi temporali concessi dalla Presidenza:

non attribuirà ulteriori spazi, per cui saranno consentiti interventi di un minuto per ciascun senatore per dichiarazione di voto, ovverosia per illustrazione di gruppi di emendamenti.

infatti, richiama un tema molto discusso in questi anni e cioè il ruolo dell'ENI nella liberalizzazione del mercato del gas in questo Paese. Ogni volta che l'ENI ci spaventa, noi ci spaventiamo e, dopo che la Commissione vota un articolo che di fatto aiuta la liberalizzazione del mercato prorogando i i tetti che scadono dal 2010 al 2015, arriva immediatamente una telefonata e qualcuno si fa carico, diligentemente, di presentare un emendamento e di sopprimere quella decisione saggia che la Commissione ha adottato. Abbiamo visto in questi giorni in televisione la *fiction* su Enrico Mattei. Tutti ricordano che Mattei è stato presentato come un coraggioso, uno che si è battuto contro le "sette sorelle" per fare in modo che l'energia in questo Paese non dipendesse

Se noi approviamo questa soppressione, nel 2010 l'ENI non avrà più alcun tetto così com'è stabilito dalla legislazione attuale introdotta nel 2000. Vi prego di valutare attentamente, perché non esiste solo l'ENI ma anche l'ENEL e l'Edison, e, come è stato ricordato nel dibattito su questo disegno di legge, l'Italia è un Paese che va solo a gas e non ha

perché, dietro la minaccia che bisogna garantire gli approvvigionamenti, i consumatori, i produttori e coloro i quali lavorano nel mercato di questo Paese vengono sottoposti ad una catena di prezzi che non è più accettabile. Prego veramente il Ministro di riflettere e di accettare il mantenimento di questo articolo.

chi vuole votare per la soppressione dell'articolo deve votare contro il mantenimento del testo e viceversa. Passiamo

su di sé la responsabilità del negoziato con l'Unione europea, per realizzare un grande investimento industriale in questo Paese.

Signor Presidente, con l'articolo 24 si vorrebbero devolvere al giudice amministrativo, in particolare al TAR del Lazio,

una disciplina processuale di questo tipo sarebbe sicuramente passibile di dichiarazione di incostituzionalità. Ricordo, peraltro, che

Ricordo ancora all'Aula, al Governo e al relatore che anche la Commissione giustizia del Senato ha già avuto modo di pronunciarsi in sede consultiva in senso negativo su questo articolo

verrebbe, infatti, ad introdurre nel nostro ordinamento giuridico processuale sostanzialmente una sorta di giudice speciale per l'intero settore energetico. Questo, ovviamente, in contraddizione palese

Inoltre, questa disposizione ci appare problematica, sotto il profilo della legittimità costituzionale nella parte in cui prevede anche un'applicazione retroattiva di questa giurisdizione esclusiva; quindi, ai procedimenti pendenti sia nella fase cautelare che nella fase di merito.

Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 24.304 (testo 2) che ha proprio lo scopo di risolvere i dubbi che sono stati in questo momento espressi dalla collega. Tentiamo di tipizzare meglio le materie specifiche che vengono devolute al TAR del Lazio nella sede di Roma e cerchiamo di definirle rigorosamente. In particolar modo, indichiamo impianti nucleari, rigassificatori, gasdotti d'importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 megawatt e le reti nazionali di gasdotti. Riteniamo, in tal modo, che la norma sia perfettamente compatibile con il quadro costituzionale.

in relazione alla parte che prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie che hanno a che fare con le procedure e i provvedimenti della pubblica amministrazione in tema di energia. Questo non appare assolutamente in linea con la giurisprudenza costituzionale ormai costante, la quale ha ripetutamente affermato la sostanziale illegittimità del ricorso al criterio di delimitazione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario fondato sul principio della ripartizione per materia. C'è poi una seconda considerazione da fare e ci rammarichiamo delle valutazioni della Lega Nord, espresse poco fa dal senatore Mazzatorta, che si è rimangiato quanto emerso all'interno della Commissione giustizia. Queste disposizioni, che fanno riferimento all'articolo 24, individuano una competenza esclusiva, per tutte le controversie concernenti il settore dell'energia, del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Questo risulta innanzitutto di dubbia legittimità costituzionale, in quanto individua una specie

propone la modifica della tabella 2 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (la finanziaria 2007, per intenderci), disponendo, in particolare, un coefficiente di incentivazione per i certificati verdi ottenuti attraverso la produzione

Presidente, sull'articolo 27-*bis* il Gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato due emendamenti che illustrerò brevemente.

che con la legge n. 6 del 1957 sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, in Italia era previsto che il concessionario del permesso di coltivazione fosse tenuto a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto calcolata sulla produzione giornaliera dei pozzi in misura che poteva raggiungere anche la percentuale del 22 per cento. Successivamente le aliquote furono unificate nella percentuale dell'8 e del 9

con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio. Si tratta di un emendamento volto a tutelare

contenuto era già presente in una mozione che il Gruppo dell'Italia dei Valori aveva presentato in data 28 gennaio 2009 e che, ovviamente, era stata respinta dall'Aula. Però proprio per l'importanza del tema, il Gruppo dell'Italia dei Valori ha voluto riproporre tale proposta oggi in questo provvedimento.

sulla questione dell'azione di classe e del risarcimento collettivo bisognerebbe fare un po' di chiarezza, perché non vorremmo che l'attuale Governo e la maggioranza,

la cronologia di questa azione collettiva. Essa venne approvata in quest'Aula per un solo voto con la finanziaria 2008 per offrire una tutela collettiva ai risparmiatori

euro coinvolgendo un milione di risparmiatori) ma anche per difendere gli utenti dei servizi bancari e le imprese che avevano subito, per oltre mezzo secolo, un'usura legalizzata denominata anatocismo (che consiste nel ricalcolo degli interessi sugli interessi). interessi sugli interessi). L'istituto dell'azione di classe significa offrire una tutela collettiva a quella classe di risparmiatori e di consumatori che possono essere raggirati da aziende eventualmente monopolistiche, che non si comportano bene e non hanno a cuore i diritti dei consumatori e neanche il rispetto delle regole del mercato.

la legittimazione ad agire concessa anche alle associazioni dei consumatori riconosciute).

Altre indicazioni sono indirizzate al versante delle procedure per chiedere una semplificazione dell'adesione dei consumatori, che eviterebbe anche la paralisi dei tribunali. La norma, nella formulazione attuale, prevede che ogni consumatore interessato depositi la documentazione in cancelleria. Questo deposito, moltiplicato per migliaia di posizioni, avrebbe l'effetto di bloccare l'operatività di molti uffici giudiziari, anche per effetto dell'accorpamento deciso sulle competenze dei tribunali. Signor Presidente, io sono abituato in quest'Aula a esprimere i concetti riguardanti la tutela dei diritti. Poi, magari,

per modificare una norma che, invece di aiutare i cittadini truffati e frodati dallo strapotere economico, oltre al danno loro anche una beffa perché, se osano promuovere nei tribunali la loro azione, essi vengono anche condannati. Cerchiamo di evitare questo e di fare davvero gli interessi dei cittadini, dei consumatori e delle famiglie, soprattutto in una fase di gravissima crisi come questa.

e le malattie. Con la *class action* come la stiamo votando noi, quelli non sono né consumatori né utenti e di conseguenza non potrebbero avvalersi dello strumento giuridico che in parte stiamo migliorando con questa norma, ma non tanto da poter far sì che quel film americano possa ripetersi anche nelle nostre aule di giustizia. Ecco perché abbiamo presentato alcuni emendamenti per sostituire

Signor Presidente vorrei pregarla, se fosse possibile, di interrompere per un quarto d'ora i lavori.

La *class action* sconta forse un peccato originale, come prima ha ricordato qualche collega; è stata approvata nell'ambito della finanziaria 2008,

sarebbe stato giusto approvarlo dopo un serio lavoro di Commissione e poi un confronto corretto in Aula, approvato attraverso lo strumento della finanziaria, sconta un peccato di approssimazione. Questa è la ragione per cui lo stesso

il mio parere favorevole all'emendamento Balboni nasce dal fatto che l'attuazione di questo provvedimento - che avrebbe dovuto subire delle modificazioni secondo le intenzioni del senatore Manzione nei primi sei mesi dell'anno 2008 - a causa della caduta del Governo e delle nuove elezioni

La legge non può che andare in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Quindi penso che l'emendamento Balboni sia particolarmente valido perché corregge una stortura pregressa. *(Applausi dal Gruppo

Con l'azione collettiva di risarcimento non introduciamo nessun reato nuovo e nessuna nuova aggravante. Non aumentiamo le pene non attribuiamo nessun nuovo diritto né nuovi poteri ai danneggiati. Non modifichiamo in nessun modo né il codice penale né le leggi fallimentari né i regolamenti della Borsa. Offriamo soltanto

televisioni, chi avrebbe tratto beneficio dalle leggi sul falso in bilancio e chi ha tratto e trarrà beneficio dai rinvii finora effettuati della legge che prevede l'azione collettiva di risarcimento.

lucido nell'analisi, come tutti gli riconosciamo, maggioranza ed opposizione, ha indicato sin dal primo momento che la causa principale della crisi è data dell'assenza delle regole, dal*deficit* di regole e di tutele. Noi, già in questa legislatura, abbiamo fatto capire come all'analisi non sono seguiti dei provvedimenti conseguenti; è iniziata con l'Alitalia e con la riduzione dei poteri dell'Antitrust. È proseguita con il recente piano casa, che nella sua prima versione prevedeva la semplificazione delle norme antisismiche,

senatore Paravia, che ha parlato di truffa. Se ci sono quelli che sono truffati due volte, sono i consumatori italiani, sono i risparmiatori che, fidandosi del sito "PattiChiari" dell'ABI, hanno investito in titoli Lehman Brothers

È assolutamente falso che, dato che non entra in vigore l'azione collettiva o di classe, oggi qualcuno, sia esso un consumatore, un contraente di un pubblico servizio o un qualsiasi cittadino danneggiato da una banca, da un'assicurazione o da un'industria, non possa far valere in giudizio i suoi diritti. Come sappiamo benissimo, qualsiasi avvocato oggi può ricevere il mandato di uno, cento, mille o un milione di clienti e proporre anche un'unica azione

Quanto alla Cirio e alla Parmalat, caro senatore Zanda, lei sa benissimo che quegli scandali sono potuti avvenire anche perché un certo Governo, presieduto da un certo Presidente del Consiglio, amico

gravissimo, di cui voi non parlate mai. Si tratta dello scandalo della Coopcostruttori, la più grande cooperativa rossa d'Italia. Parliamo di un miliardo di euro che Donigaglia, principale finanziatore di Botteghe oscure, ha fatto sparire, sottraendoli ai pensionati e alla povera gente.

Poiché la *class action* è una norma comunque rivoluzionaria nel nostro ordinamento, mi sembra logico e ragionevole che venga applicata ai casi futuri, ai nuovi illeciti...

soppressivo dell'articolo 30-*bis*, perché siamo profondamente interessati a che tutti i soggetti che siano stati lesi a destra, a sinistra e al centro, siano nelle condizioni di poter esercitare una volta per tutte l'azione collettiva a tutela dei propri diritti che, per definizione, non possono essere tutelati individualmente. Come è noto, infatti, nessuno di noi ha questa grande dimestichezza con tutte le clausole contrattuali espressamente sottoscritte, la cui dimensione tipografica è al di sotto del micron,

sull'azione collettiva, la *classaction*. Il ministro Tremonti dice che non parla l'inglese; non è un demerito, per carità di Dio, ma è evidente che il tema è

Se, viceversa, le imprese americane o straniere vengono in Italia, i consumatori italiani non hanno alcuna possibilità di esercitare un controllo diretto e avere una tutela collettiva di una serie di diritti e di interessi giuridicamente Questo è il tema del confronto alla concentrazione imprenditoriale, anche nel nostro Paese, attraverso le multinazionali, le quali operano in maniera differenziata a seconda del regime giuridico che si trovano di fronte. Se noi non adeguiamo le regole del nostro sistema sotto il profilo della tutela dei consumatori, ci ritroviamo a fare una cortesia non alle imprese italiane, ma a quelle imprese che hanno un regime di maggior favore in danno dei consumatori nel nostro Paese. Questa è la questione rispetto alla quale la politica del rinvio e la politica della irretroattività non fanno altro (al di là del merito della singola questione, se possa essere più o meno opportuna, se le vicende relative alla disciplina dei cosiddetti diritti identici sia utile a far esperire l'azione collettiva o, viceversa, metta i consumatori nelle condizioni di non poterla esperire)

a operare con un regime differenziato nel nostro Paese perché hanno un'isola felice, in cui possono operare senza avere alcun controllo collettivo da parte dell'utente principale, del soggetto protagonista del libero mercato - di cui tutti ci riempiamo la bocca - che è il cittadino consumatore e le famiglie italiane. Questa è la responsabilità grave che vi state assumendo con l'ennesima modifica della disciplina sulla *classaction*,con il rinvio della sua entrata in vigore e con la previsione della irretroattività della stessa disciplina, misure che colpiscono peraltro, come è stato già detto, i piccoli azionisti che hanno creduto nell'azionariato diffuso rispetto alle nostre imprese italiane. Questo è il dato politico di cui vi dovete assumere la responsabilità

del mio Gruppo, espressa dal senatore Zanda. Senatore Balboni, la differenza tra il diritto sostanziale e il diritto all'azione credo che l'abbiamo chiara tutti in quest'Aula, o almeno quasi tutti, così come abbiamo assolutamente chiare le vicende

Adesso, le voglio raccontare una vicenda, che non è un aneddoto, ma un pezzo di storia parlamentare, proprio perché lei continua a ragionare sulla rivoluzione introdotta dalla *class action* e sul fatto che le rivoluzioni bisogna un po' ritardarle. È una rivoluzione infinita: di *class-action* si parla nelle Aule della Camera e del Senato, a mia memoria, almeno da 12 anni. La vicenda risale al Governo Berlusconi.

Allora la competenza per chi volesse chiedere il risarcimento del danno relativo ai questi 47 euro di premio in più pagati era del giudice di pace. Come tutti i cittadini e tutti i consumatori sanno, dinanzi al giudice di pace si va senza avvocato e soprattutto non si può, quando si tratti di una somma quale quella che era dalle richieste dei consumatori, ricorrere in appello. Il Governo Berlusconi si convocò e con grande attenzione alle ragioni delle grandi assicurazioni italiane - tutte tutte - decise di varare immediatamente un decreto perché per quei 47 euro la competenza venisse spostata dinanzi al tribunale, con la conseguenza che occorreva munirsi di un difensore, quindi pagare un avvocato, e che si andava incontro alla possibilità di ricorso in appello, che certamente le grandi lobby assicurative avrebbero fatto. Il risultato fu che centinaia di migliaia di cittadini italiani rinunciarono all'azione perché per 47 euro non valeva la pena di far valere il proprio diritto.

e che ovviamente avevano lo stesso identico interesse di altre compagnie che facevano riferimento ad altri soggetti. Da lì partì con rinnovata lena il nostro lavoro sulla *class action*. Ho dovuto approfittare del voto in dissenso per poter raccontare questo pezzo della storia italiana e per mettere un punto a questo affresco sulla rivoluzione che, a vostro avviso, se arriva oggi è troppo presto. Meglio che arrivi tra 10 anni, o forse mai più, tanto gli interessi

**Il Senato non approva.**